del rispetto delle identità di genere sia compreso negli obiettivi nazionali di istruzione, si fa presente che la materia è trattata nell'ambito dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», introdotto con la legge n. 169 del 2008, e nell'ambito dei progetti educativi sul problema della legalità, attivi presso le scuole di ogni ordine e grado. Si è consapevoli, peraltro, che il fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica ha assunto, negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupati per una società civile. Per questa ragione non si mancherà, in occasione di una revisione delle linee guida riguardanti il citato insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», di dare ancora maggiore rilievo al tema dell'educazione all'uguaglianza, con particolare riferimento alla prevenzione delle discriminazioni e dei sessismi, atteggiamenti suscettibili di degenerare in meccanismi patologici di violenze nei confronti delle donne. Si segnala che sono allo studio specifici percorsi di insegnamento, da introdurre all'interno dell'educazione alla cittadinanza, fin dall'inizio della scolarizzazione degli allievi. Si ritiene poi che i temi in discussione dovrebbero anche caratterizzare la pianificazione di attività formative indirizzate ai docenti, ai dirigenti scolastici e al personale ATA. Le iniziative in tal senso potrebbero realizzarsi in *partnership* con i Ministeri delegati per le pari opportunità, le politiche giovanili, l'integrazione, il lavoro e politiche sociali e la salute, con il coinvolgimento delle associazioni e i movimenti impegnati in concrete azioni di sostegno alle vittime di violenza. L'apporto di coloro che conoscono i danni e le ricadute del fenomeno potrebbe infatti costituire un valore aggiunto per informare, in particolare i docenti e i dirigenti scolastici, sui fattori che possono influire sul successo formativo degli alunni che vivono in contesti familiari a rischio. In merito al recepimento nei libri di testo delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione predisposto secondo il progetto POLITE si ricorda si ricorda che, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica dovrà adeguare i testi delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai contenuti delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo, emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012. In questa prospettiva, si rassicura che il Ministero promuoverà una specifica opera di sensibilizzazione verso gli operatori editoriali al fine di favorire, nel rispetto della libertà di stampa costituzionalmente garantita ad autori ed editori, l'adozione e la diffusione del citato progetto.

Benissimo, sono fondamentali le azioni di formazione. Soprattutto potrebbero essere inserite

È fondamentale che anche nei libri di testo venga recepito quel codice POLITE su cui l'associazione degli editori di libri di testo scolastici ha lavorato assieme assieme al Ministero. È importante sottolineare che è a scuola che possiamo davvero educare nuove generazioni di uomini e donne rispettosi delle differenze e delle libertà libertà individuali. È a scuola che possiamo insegnare alle ragazze che è solo con lo studio e con il lavoro che si diventa davvero libere ed è a scuola che possiamo insegnare alle nostre figlie anche a crescere nella consapevolezza che uno schiaffo è uno schiaffo e non è mai amore. Pertanto, la ringraziamo per questo impegno. Questo Parlamento, e in particolare la 7a Commissione, vigilerà sull'operato assieme al vasto mondo dell'associazionismo femminile, che è impegnato - appunto - a promuovere la differenza di genere: una vera cultura della differenza di genere.

Signora Presidente, si ricorda che la programmazione e l'attuazione di iniziative per il contrasto alle discriminazioni sono state avviate già a partire dal 2007, con la direttiva n. 16 del 5 febbraio, contenente «Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo». Rispetto al più specifico problema dell'omofobia, diverse sono le iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno. Già nell'atto parlamentare viene fatto riferimento alla «Settimana contro la violenza», che a partire dal 2010 si tiene ogni anno, dall'11 al 17 ottobre, nelle scuole di ogni ordine e grado, e alla «Giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia», che si svolge il 17 maggio di ogni anno. In queste occasioni gli istituti scolastici realizzano attività educative che consistono in azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, sulla prevenzione della violenza, dell'intolleranza razziale, religiosa e di genere, nonché di ogni forma e causa di discriminazione. Durante la settimana contro la violenza, gli studenti hanno modo di confrontarsi con esperti e operatori delle forze di polizia, al fine di acquisire una maggiore conoscenza degli strumenti legislativi vigenti nel nostro Paese. Sempre a proposito delle iniziative realizzate in argomento, si ricorda l'istituzione, presso la direzione generale dello studente del Ministero dell'istruzione, del servizio di assistenza telefonica tramite il numero verde per il bullismo,

chiamato a collaborare con la citata direzione generale dello studente per realizzare occasioni di incontro e condivisione tra alunni, famiglie e operatori del settore, affinché lo scambio delle diverse esperienze professionali sia di incentivo per la crescita morale e per l'azione educativa degli studenti. Per una migliore condivisione delle esperienze e delle campagne attuate dagli uffici scolastici regionali, il Ministero ha anche realizzato un portale «www.noisiamopari.it» che dà evidenza delle iniziative positive sul tema, con l'intento di condividere i programmi a carattere educativo che i *partner* della rete svolgono anche a livello locale. orientamento sessuale e identità di genere), che nasce nel 2006 su iniziativa di un gruppo di amministrazioni locali e regionali e si propone di favorire politiche di parità tra sessi, rispetto dell'orientamento sessuale e dell'identità dell'identità di genere, nonché di diffondere buone prassi sul territorio nazionale. Quanto alla formazione rivolta al personale scolastico, i temi in discussione dovrebbero senza dubbio caratterizzare la pianificazione delle attività formative. Come già ricordato, si ritiene opportuno che siano realizzate iniziative in collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte, nonché con le associazioni e i movimenti impegnati a fornire supporto alle vittime di violenza. Tra le iniziative già intraprese, si ricorda la *partnership* avviata dalla direzione generale per il personale scolastico con l'Osservatorio nazionale bullismo e *doping*, un'associazione senza scopo di lucro che mira a realizzare sull'intero territorio nazionale campagne di comunicazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *doping*, ritenendo tali fenomeni fattori di condizionamento del comportamento e dello stile di vita della popolazione giovanile. Con decreto direttoriale n. 35 del 21 giugno 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro nazionale paritetico con il compito di progettare e pianificare azioni di sensibilizzazione, di informazione e di formazione, rivolte a tutte le componenti scolastiche, per promuovere iniziative ed eventi che favoriscano la riflessione sul valore educativo della pratica sportiva e sui corretti stili di vita da assumere per una consapevole partecipazione democratica alla vita della comunità. È in corso di sottoscrizione anche un protocollo d'intesa di durata triennale attraverso il quale realizzare attività formative incentrate sul valore educativo dei percorsi professionali compiuti da personaggi del mondo della cultura e dello sport, i quali abbiano perseguito i propri obiettivi con modalità e valori che possono essere di esempio per gli studenti. [LO

debbano senza dubbio caratterizzare le azioni di pianificazione formativa delle scuole italiane.

di dirigenti, insegnanti ed educatrici che si trovano a confrontarsi con il problema. Mi riferisco alla presenza nelle scuole di bambini che crescono in famiglie omogenitoriali, ossia con due mamme o con due papà, e che per questo

se e come il Governo, in particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, intenda affrontarlo. Rispetto alla questione della partecipazione del Ministero dell'istruzione alla strategia nazionale

ritengo molto importante che gli obiettivi e gli intendimenti qui espressi possano essere in qualche modo condivisi

realtà, adeguata agli *standard* umanitari, poteva essere garantita a coloro che dovevano essere identificati e poi espulsi. Cosa succede? Quando arriva il Governo Monti, il Ministero dell'interno decide che l'importo *pro capite*, che per i centri piccoli era di circa 70 euro,

che è andato in pensione un mese fa. Detto prefetto, quand'era a Siracusa, aveva dato a trattativa privata alla cooperativa "L'Oasi" il centro di Siracusa. Chiaramente

che aveva ottenuto un finanziamento per il centro immigrati di Cassibile, ma la cattiva gestione del centro aveva costretto il Comune di Siracusa ad aprire un contenzioso per mancanza di rendicontazione. Poi c'era stato il rinvio a giudizio di Marco Bianca, quindi tutto un pregresso di cattiva gestione dei centri. A Modena c'è stata una gara:

e che pagavano i bonifici? Per esempio, il signor Emanuele Midolo è stato condannato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa, il 19 ottobre 2011, alla pena di quattro mesi di reclusione per i reati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e di falsità materiale commessa da privato. La condanna è stata definita per patteggiamento, quindi è definitiva:

li ha pagati con mesi di ritardo), in una situazione in cui gli enti locali, i sindacati, le organizzazioni umanitarie, che ripetutamente in questi mesi si sono interessati del problema, hanno fatto relazioni raccapriccianti

garantire quel trattamento che pure nei capitolati è previsto, quindi la mediazione culturale, l'assistenza medica e così

tutto il meccanismo degli accordi internazionali è una risposta intelligente a un fenomeno esistente. Io sono per l'integrazione, come ho detto un milione di volte. Facciamo ogni anno feste etniche con tutte le etnie, dai filippini ai senegalesi, dai ghanesi ai cinesi, sono tutti amici. Ma

Ma questa scelta non la pagherebbe il Governo, bensì la gente normale, specialmente chi vive non nei quartieri alti ma in quelli dove si convive con queste forme di criminalità.

Vuol dire che torneremo con un'altra interpellanza dopo aver preso altre informazioni. Ma poiché mi sembra che quello che abbiamo scritto e documentato, fin dall'inizio, sia un po' surreale, rimane sempre la domanda: cosa ci vengono fare a Milano, a Modena e a Bologna cooperative che, fin dall'inizio, non sono in grado di gestire strutture simili? Cosa ottengono in cambio dei 29 euro *pro capite*? Che finalità si pongono? Perché vengono a lavorare al Nord? Perché, abituata ad uno *standard* di servizi di un certo tipo, la nostra società deve

in questa occasione, felice della presenza di un Sottosegretario che ha approfondito la materia, ci fosse la possibilità, non di una risposta interlocutoria, banale o burocratica, ma di una risposta che desse un contributo a risolvere questo problema. Ricordo anche le difficoltà dei dipendenti,

interrogazioni al Governo e di sollevare il problema, non può fare. Quindi, mi aspetto questa mattina una risposta che dia almeno l'avvio alla soluzione del problema.

Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, anch'io proverò a documentare e circostanziare la questione cui ha già accennato il collega Giovanardi. L'interpellanza con procedimento abbreviato che ho presentato assieme ad altri colleghi sulla grave situazione dei centri per l'identificazione e l'espulsione di Modena, Trapani e Bologna, fa seguito alle interrogazioni che le colleghe Orrù e Puglisi, il collega Lo Giudice ed io avevamo già presentato in merito a ognuno dei suddetti centri. I fatti accaduti nell'ultimo mese, soprattutto presso il CIE di Modena, sono talmente gravi da richiedere una risposta immediata e chiara da parte del Governo affinché non si ripetano più situazioni di oggettiva e, ahimè, prevedibile insostenibilità nella gestione di strutture come queste. Ricordo, infatti, che tutti e tre i CIE sono gestiti dalla medesima cooperativa, "L'Oasi" di Siracusa, che si è aggiudicata la gestione dei centri in presenza di criteri di valutazione difformi e orientati al massimo ribasso. Ciò si è verificato, ad esempio, nel maggio 2012, quando la prefettura di Bologna mise a bando la gestione del CIE di via Mattei con il criterio del massimo ribasso e la base d'asta fu di 30 euro al giorno per persona: la cooperativa "L'Oasi" si aggiudicò la gestione della struttura con un'offerta di 28,5 euro a persona a persona al giorno, a fronte dei 69 euro corrisposti al precedente gestore. La vicenda del CIE di Modena è in questo senso emblematica. Dal 2007 e fino al 30 giugno 2012, il CIE della città è stato gestito in appalto dalla Confraternita della Misericordia, che riceveva dalla prefettura di Modena 75 euro al giorno per trattenuto. Il 15 febbraio 2012 è stato pubblicato il bando per l'affidamento della gestione, che ha stabilito come base d'asta la quota di 30 euro al giorno per trattenuto, con presentazione dell'offerta entro il 15 marzo 2012 ed aggiudicazione prevista attraverso il criterio del massimo ribasso. La CGIL di Modena ha da subito sostenuto, assieme a tante altre forze, forze, che la base d'asta non era sufficiente a garantire il rispetto di quanto previsto nel capitolato ed al tempo stesso il rispetto delle leggi, delle norme e dei contratti e che il criterio del massimo ribasso finiva di fatto con l'impedire la partecipazione ai bandi proprio a quelle imprese che offrono maggiori garanzie di affidabilità. L'unica offerta presentata è stata quella della Confraternita della Misericordia di Modena che, tuttavia, non è stata presa in considerazione perché superiore alla base d'asta stabilita. La prefettura di Modena ha quindi attivato una procedura ristretta, tramite inviti a presentare offerte, alla quale si è presentata solamente la ho citato, che si è aggiudicata la gestione con un ribasso del 3 per cento rispetto alla base d'asta, e quindi a 29,1 euro al giorno per trattenuto, subentrando così, dal 1° luglio 2012, nella gestione. Sin dall'inizio della gestione, i dipendenti del consorzio hanno avuto difficoltà a ricevere i propri stipendi, e solo il pagamento di questi da parte della prefettura, ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile, ha consentito, a più riprese, di sbloccare la situazione. Infatti, mentre lo stipendio di luglio 2012 è stato pagato in ritardo, quelli di settembre ed ottobre non sono stati pagati. Dopo varie promesse disattese da parte del consorzio, la Funzione pubblica-CGIL ha proclamato uno sciopero per il 10 dicembre 2012 pochi giorni prima di questo gli stipendi sono stati pagati, a seguito di un interessamento della prefettura di Modena. Il 25 gennaio 2013, è stato proclamato un nuovo sciopero. Il giorno prima, il ministro dell'interno *pro tempore* Cancellieri, in visita a Modena, aveva annunciato che i lavoratori sarebbero stati pagati entro pochi giorni.

svoltesi tra febbraio e marzo, la prefettura si è fatta poi interamente carico del pagamento delle mensilità di dicembre, della tredicesima mensilità 2012 e di quelle di gennaio e febbraio 2013. La stessa situazione si è ripetuta nei mesi successivi. successivi. Dall'inizio della gestione, quindi, di 13 mensilità soltanto una è stata pagata regolarmente ai lavoratori; le altre, in ritardo, sono state erogate dalla prefettura, ma dal mese di maggio i lavoratori del centro non ricevono alcuna retribuzione. Inoltre, va sottolineato l'avvicendamento di ben quattro direttori, talvolta per il mancato pagamento del loro stesso stipendio, ciò che ha reso impossibile ogni stabile programmazione interna delle attività e ogni efficace relazione con tutti i soggetti coinvolti, dentro il centro e fuori da esso. Nella giornata di sabato 6 luglio, a fronte del permanere e dell'acutizzarsi dei problemi, la CGIL di Modena ha proclamato altri sei giorni di sciopero consecutivi per i lavoratori che operano nel centro. Tale fatto, oltre a rimarcare una volta di più l'insostenibilità della situazione, avrebbe rappresentato senz'altro un delicatissimo problema per la sicurezza del centro stesso, sapendo quali ripercussioni avrebbe potuto avere sulla vita dei trattenuti, allora 36, una sospensione dei servizi, soprattutto all'avvio del periodo del Ramadan. Ancora una volta, solo l'intervento della prefettura ha determinato una iniziale sospensione dello sciopero, a fronte di impegni assunti dalla stessa nei confronti dei lavoratori. Lo sciopero dei lavoratori, prorogato, ha comunque avuto inizio solo martedì 23 luglio e si protrarrà sino a domenica 28 luglio. Come è noto, uno sciopero di tale lunghezza non è ammesso dal legislatore, che ne consente una durata massima di 48 ore. Per tale motivo, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha aperto un procedimento per inadempienza nei confronti della Funzione pubblica-CGIL di Modena. Tale procedimento è stato tuttavia subito archiviato dalla Commissione, che ha optato per il non luogo a provvedere né verso i lavoratori né verso il sindacato, dichiarando la presenza di una condizione di «eccezione di inadempimento». La Commissione ha cioè riconosciuto le inadempienze del consorzio talmente gravi da ritenere legittima da parte dei lavoratori l'adesione ad uno sciopero più esteso delle 48 ore consentite. Tale decisione della Commissione di riconoscere una eccezione di inadempimento si è peraltro verificata in rari, e veramente gravi, casi, dal 1990 ad oggi. Ma l'azione intrapresa dalla Commissione di garanzia è andata anche oltre. L'Autorità ha infatti deciso di avviare un'indagine conoscitiva sui reali motivi che impediscono al consorzio di corrispondere regolarmente le mensilità ai propri dipendenti. La lettera dell'Autorità al consorzio è stata inviata il 10 luglio scorso, ma al momento non sono state date ancora risposte. Questa circostanza, signor Sottosegretario, non è affatto irrilevante: si tratta del primo caso in assoluto in cui la Commissione di garanzia si muove al fine di accertare delle responsabilità in capo ad amministrazioni che contribuiscono ad aumentare il livello del conflitto anziché attenuarlo. possiamo ben immaginare che questa prassi inaugurata dalla Commissione sulla vicenda del CIE di Modena si ripeterà sempre più spesso nei confronti delle sempre più frequenti situazioni di mancata corresponsione degli stipendi ai lavoratori. Peraltro, dopo avere incontrato a più riprese Funzione pubblica-CGIL e i lavoratori, nella giornata di sabato 6 luglio ho personalmente effettuato, a sorpresa, assieme agli onorevoli Baruffi e Patriarca, una lunga visita una lunga visita al centro, in cui abbiamo potuto riscontrare direttamente le carenze lamentate da più parti, una qualità decisamente inadeguata delle strutture, una condizione igienico-sanitaria insostenibile e un'esasperazione dei trattenuti derivante anche da questo stato di cose, che diventa ancor più insostenibile nei mesi estivi dell'anno. Giovedì 11 luglio la Guardia di finanza di Modena ha poi perquisito, su mandato del pubblico ministero Marco Niccolini, gli uffici del consorzio all'interno del centro, per far luce su come sia sostenibile per il suddetto gestire una struttura con soli 29,1 euro al giorno per trattenuto. la situazione al CIE di Modena è poi precipitata nell'ultima settimana, a seguito dello scoppiare di alcune rivolte da parte degli ospiti, che hanno provocato danni stimati dalla prefettura tra i 50.000 e i 70.000 euro e l'arresto di nove cittadini tunisini. Lunedì 22 luglio si è svolta l'udienza davanti al gip, a seguito della quale è stata disposta la permanenza in carcere per tre di questi e il rilascio con obbligo di dimora per i restanti sei. Tuttavia, le motivazioni della rivolta dichiarate dai nove cittadini tunisini sono risultate talmente gravi e riconducibili alla presenza di condizioni igieniche nel centro estremamente precarie che il gip ha rimandato gli atti alla procura per la verifica di eventuali reati a carico del gestore e all'AUSL di Modena, prospettando un interessamento diretto anche del sindaco della città per motivi di sanità pubblica. La situazione drammatica in cui versa il CIE è stata confermata anche dal segretario nazionale del SIULP Felice Romano, che alcuni giorni fa ha dichiarato in una nota come il centro sia ormai «un *lager* per immigrati e poliziotti». Un comportamento analogo a quello tenuto verso i lavoratori del CIE di Modena la cooperativa di Siracusa lo ha mostrato anche verso quelli operanti nelle sedi di Trapani e Bologna. A Trapani, nonostante le irregolarità rilevate dagli ispettori del lavoro nella gestione del CIE, il 16 gennaio 2013 il consorzio "L'Oasi" espresse l'intenzione di assumere 15 nuovi dipendenti, pur non riuscendo a pagare con regolarità gli stipendi agli oltre 50 lavoratori già in servizio presso la struttura. A Bologna, sin dall'avvio della nuova gestione, il consorzio assegnatario non ha pagato gli stipendi ai 29 dipendenti Le situazioni descritte richiedono pertanto un intervento urgente da parte del Governo, cui chiediamo, anzitutto, quali azioni di propria competenza intenda adottare per garantire i lavoratori e le forze dell'ordine che operano presso i CIE se non ritenga che l'adozione della modalità di aggiudicazione della gara secondo il meccanismo del massimo ribasso si sia rivelata inadeguata alla gestione dei suddetti centri. Chiediamo inoltre se non ritenga che vi siano state da parte dello stesso consorzio gravi, ripetute e sistematiche violazioni della convenzione, tali da comportare la revoca della stessa. Infine, le chiediamo, signor Sottosegretario, se non ritenga utile avviare una seria riflessione sull'utilità dei centri di identificazione ed espulsione per valutare l'eventuale inadeguatezza dei CIE rispetto all'obiettivo di ridurre l'immigrazione irregolare,

arrivare subito al cuore del problema. Il cuore del problema è indiscutibilmente la base d'asta fissata (ovviamente non da questo Governo, ma

una forma di distorsione nell'accesso alla convenzione, perché molto spesso le gare vanno deserte, e altrettanto spesso vi è un solo concorrente che fa la proposta e inevitabilmente si aggiudica l'appalto:

nei confronti della prefettura di Modena, perché così non è. Infatti, tenuto conto che la risoluzione del contratto compete comunque alla prefettura del posto e non al Ministero, si stanno valutando tutte le inadempienze che sono state registrate e che ‑ ahimè ‑ ormai cominciano ad essere tante (anche se interferiscono con l'esistenza di processi penali, che hanno visto coinvolti gli interni e i gestori del centro), al fine di verificare se sussistono gli estremi per poter risolvere il rapporto con la cooperativa "L'Oasi". Questo, da un punto di vista strettamente limitato al rapporto tra il CIE di Modena e la cooperativa Più in generale, tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui versiamo attualmente, credo si possa immaginare di intervenire su due fronti.

Ovviamente, ciò va fatto compatibilmente con le risorse economiche che si riescono a trovare, altrimenti, se non si potrà incidere sulle risorse economiche o se non si potrà ottenere sufficienti risorse economiche, bisognerà immaginare di lavorare sull'elenco dei servizi, cioè ridurre i servizi che possono essere prestati, in maniera da rendere competitiva la risorsa economica, se rimane scarsa come quella che viene fornita oggi. L'altro intervento, che credo sia in linea con quanto diceva lei, senatore Giovanardi, potrebbe essere quello di diversificare i prezzi di accesso, con riferimento al numero delle persone presenti nei centri, in maniera tale che che non ci sia un unico contratto in tutt'Italia che prescinde dalle possibili economie di scala che la presenza di un numero di persone sufficientemente elevato può consentire, rispetto al centro di minori dimensioni. Questi, a risorse invariate - perché, evidentemente, se riuscissimo a recuperare maggiori risorse il problema si risolverebbe di per sé - potrebbero essere due degli aspetti sui quali non faccio difficoltà a dire che il Governo si impegna ad intervenire.

in un certo senso, la permanenza nel CIE è psicologicamente molto più afflittiva rispetto a quella in carcere, quindi può dare luogo a fenomeni come quelli che si sono verificati a Modena, per l'ottima ragione che la pena ha un inizio e una fine che sono scanditi da un provvedimento giudiziale e il soggetto che deve affrontarla sa esattamente il percorso che deve

senza che sia stato «generalizzato» effettivamente, ciò provoca probabilmente uno stato d'animo che può influire sulle condizioni complessive.

Allora, dal punto di vista amministrativo, gli interventi che mi sono venuti in mente sono i primi due che vi ho rappresentato; dal punto di vista normativo il percorso, ovviamente, è più lungo e necessita di un supporto, anche parlamentare, assai consistente. Vedremo se questo Governo sarà in grado di procacciarselo.

Apprezzo molto la sua iniziativa nel voler apportare modifiche sia a livello normativo che amministrativo, però innanzitutto ci dovrebbe essere un intervento amministrativo, che è quello più veloce e forse urgente,

ripeto - è assolutamente urgente che si ripensi la modalità di assegnazione di questi centri, perché ogni giorno che passa a 29 euro a persona significa violazione dei diritti umani fondamentali.

che, rispetto agli obiettivi che si era posto, ha dimostrato tutti i suoi limiti.

da parte delle autorità competenti. Rimane sicuramente qualcosa da verificare, anche per impedire che in futuro accadano nuovamente situazioni

chiusi e non possono quindi neanche corrispondere alle esigenze per le quali sono stati creati. Occorre trovare un meccanismo prima che, come al solito, intervenga la procura della Repubblica con arresti; è opportuno che siano le autorità competenti a provvedere, come a Bologna, alla revoca di questa convenzione. Non c'è sempre bisogno che arrivi l'autorità giudiziaria alla fine, quando le cose sono ormai evidenti; dovrebbe essere l'Esecutivo e le sue strutture periferiche, come a Bologna, a

ma come, questa persona è irregolare, ha avuto il decreto d'espulsione ed è in giro libera di ammazzare, rapinare e stuprare? Certo: se non c'è un luogo dove trattenerla in attesa dell'espulsione, c'è il pericolo reale che accadano fatti di questo tipo, che l'ordinamento deve evitare.

è mica il posto in cui la Polizia e i Carabinieri per fare statistica devono andare a vedere se c'è la badante russa o quella ucraina che magari hanno il visto scaduto.

domande, perché ha parlato di distorsione nel momento in cui si ragiona su criteri di assegnazione come quelli che abbiamo citato

di fare presto, perché la situazione, oltre che grave, non è più rinviabile. Credo che anche dai dati che ho cercato di portare, in aggiunta a quelli di cui lei sicuramente disponeva,

ancorché sul lato politico-normativo dell'idea di riforma delle strutture dei CIE.

una collaborazione per aprire questa discussione in modo ampio, franco e complessivo, troverà sicuramente nei senatori

effettuate durante le ultime elezioni amministrative, con particolare riferimento ai Comuni di Maddaloni e Marcianise, in provincia di Caserta. In effetti, in occasione delle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio scorsi, la prefettura di Caserta ha proposto alle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale la sottoscrizione di un protocollo riguardante il quadro complessivo delle regole che disciplinano lo svolgimento della propaganda elettorale. Con il predetto atto, al quale hanno aderito, unitamente ai rappresentanti delle forze dell'ordine, tutti i partiti rappresentati in Parlamento, oltre a numerose liste civiche, nel richiamare l'attenzione sull'attività di affissione dei manifesti elettorali, si è anche sottolineato l'obbligo di utilizzazione esclusiva degli spazi appositamente riservati, nonché il dovere delle amministrazioni comunali di provvedere alla rimozione dei manifesti abusivi o affissi al di fuori degli spazi autorizzati. Al riguardo i comandi della polizia municipale di Maddaloni e Marcianise si sono tempestivamente attivati per reprimere tale fenomeno. Sono stati infatti accertati numerosi illeciti amministrativi nei confronti di committenti e candidati alle elezioni e, pertanto, attivate le conseguenti operazioni di oscuramento. In particolare, nel Comune di Maddaloni sono stati adottati 226 verbali di illecito amministrativo, con l'oscuramento di circa 550 manifesti abusivi, mentre nel Comune di Marcianise gli accertamenti sono stati 44. Va sottolineato che già nei primi giorni della campagna elettorale, non appena il fenomeno si è manifestato, sono state prontamente adottate iniziative di contrasto, anche grazie all'ausilio delle forze dell'ordine, che nel Comune di Maddaloni hanno contestato circa 250 violazioni. Nell'interrogazione si fa riferimento alla richiesta rivolta da uno dei candidati alla carica di sindaco al competente ufficio di Maddaloni affinché lo stesso provvedesse all'affissione Al riguardo l'ente locale ha precisato che, in base al regolamento comunale, tale attività non è mai stata gestita dai dipendenti del servizio affissioni. Relativamente agli esposti sugli abusi commessi in materia di propaganda elettorale, le forze dell'ordine hanno tempestivamente informato l'autorità giudiziaria. In merito, infine, ai presunti episodi di voto di scambio, la prefettura di Caserta ha provveduto,

ad alta infiltrazione camorristica e mafiosa, però venivano segnalati soprattutto episodi di voti di scambio e di corruzione elettorale, talvolta documentati, anche in quest'ultima campagna elettorale, da *blog* locali, da emittenti locali, anche dai singoli candidati, che avrebbero meritato ben altra attenzione e ben altra preoccupazione da parte dell'ufficio territoriale di Governo, presso il quale io stessa

la commistione tra la semplice - per modo di dire - corruzione elettorale e il controllo del voto per altre finalità (cioè quelle mafiose) è talmente labile e sottile che forse sarebbe valsa la pena di ma da parte di chi era stato interessato per una vigilanza più attenta. Stiamo anche parlando di una zona (di due Comuni, che poi sono quelli che ricadono nell'area industriale sostanzialmente) dove già in un passato recentissimo si è accertato che a gestire la campagna di affissioni sono persone che fanno riferimento direttamente al maggiore *clan* camorristico della zona, appunto il *clan* dei casalesi, controllati direttamente da esponenti di primo piano. Quindi, una sollecitazione del Governo agli organismi territoriali e una maggiore vigilanza specifica su questi temi sarebbero gradite.

*(PD)*. Signora Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione su una situazione che riguarda il mio territorio, la provincia di Trapani, ma che ha ripercussioni su tutto il territorio nazionale in termini di mancata ricaduta economica legata al turismo della mia Regione e dell'Italia, oltre che sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri. Si tratta dell'interruzione della tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo. In particolare, il tratto che collega Trapani ad Alcamo, a seguito di un cedimento strutturale, è stato chiuso al traffico dal 25 febbraio scorso. Da febbraio ad oggi la tratta non è mai stata riaperta e RFI, che gestisce per conto di Ferrovie dello Stato SpA l'intera rete ferroviaria italiana, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dall'11 agosto prossimo. La tratta ferroviaria in questione è strategica per la mia Provincia, in quanto la allaccia all'aeroporto di Birgi e, soprattutto, mette in collegamento i due aeroporti della Sicilia occidentale. È una via cruciale per lo sviluppo del territorio che necessita di potenziamento, non di interruzioni e dismissioni, e che però, poiché i problemi della linea sono di tipo strutturale, sembra essere stata dimenticata dal Programma infrastrutture strategiche emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aprile scorso. Finora il percorso è stato assicurato da un servizio sostitutivo effettuato in pullman, ma anche questo sembrerebbe a rischio (forse rimarrà attivo soltanto per un breve periodo). In pratica, da metà agosto si potrà andare a Trapani da Palermo con il treno solo attraverso via Castelvetrano, impiegandoci ben cinque ore. Richiamo l'attenzione del Governo, in quanto già da tempo è stata rivolta dai sindacati del settore e dalla popolazione locale coinvolta la richiesta - più volte reiterata non solo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche al Presidente della Regione e ad altri organi che potrebbero essere interessati - di prevedere il ripristino della tratta in questione che, come dicevo all'inizio, collega strategicamente i due aeroporti. aeroporti. Con questo intervento, preannuncio che presenterò un'interrogazione al Governo per conoscere gli effettivi orientamenti sulla tratta in questione.